Onorevoli colleghi, in esito alla conclusione, da parte dell’8ª Commissione permanente, dell’esame dei disegni di legge recanti disposizioni in materia di sicurezza stradale, il Presidente della Commissione medesima ha trasmesso ieri sera alla Presidenza la richiesta di riassegnazione dei predetti provvedimenti in sede redigente, con l’assenso dei rappresentanti dei Gruppi. Non appena pervenuto l’assenso del Governo, i disegni di legge nn. 1720 e connessi saranno riassegnati in sede redigente alla 8ª Commissione permanente, che efin d’ora autorizzata a convocarsi. E[ ]inoltre autorizzata a convocarsi, per i pareri, la Commissione bilancio. La discussione dei disegni di legge in questione – ove conclusi in Commissione – avra` luogo in Assemblea nella seduta pomeridiana di oggi, nel corso della quale saranno esaminate anche ratifiche di accordi internazionali. Pertanto, la mattinata potra` essere utilizzata anche dalle altre Commissioni permanenti per lo svolgimento dei propri lavori.